Signor Presidente, ringrazio l'onorevole interrogante per la questione posta con tempestività. Devo dire che, in riferimento all'episodio che ha coinvolto il cronista dell'emittente televisiva "Eleven Sports" (una piattaforma televisiva che trasmette eventi sportivi, in particolare calcistici), fortunatamente abbiamo recuperato un increscioso incidente. Ricordo che, durante la telecronaca della partita del campionato di Serie C Trento-Vicenza, parlando del giocatore di colore del Vicenza Greco, equivocandone il nome, lo ha ribattezzato "Negro". Al riguardo comunque ricordo - come già detto - che preliminarmente lo stesso telecronista, resosi immediatamente conto dell'imperdonabile *lapsus*, si è scusato in diretta e che l'emittente televisiva "Eleven Sports", dopo aver prontamente sospeso in via precauzionale il telecronista, ha emesso un comunicato, reso noto dal Vicenza calcio, in cui si afferma: «Nonostante l'accaduto sia da ricondurre ad una gravissima leggerezza da parte del collaboratore, ci sentiamo di affermare che dietro a questo episodio non si cela alcuno sfondo razzista e non sarebbe corretto considerarlo sotto altra veste, lontana sia dal *modus operandi* di Eleven Sports sia da quello del commentatore stesso». Resta inteso che, riguardo alle iniziative invocate dall'interrogante, si rappresenta che i compiti di vigilanza cui fa riferimento sono da ascrivere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale ha il potere sanzionatorio di irrogare diffide e sanzioni. In particolare, nel 2019 l'Autorità ha adottato la delibera n. 157, che contiene le disposizioni cui devono adeguarsi cui devono adeguarsi i fornitori di servizi dei media audiovisivi e radiofonici soggetti alla giurisdizione italiana, per assicurare il rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e contrasto alle espressioni di odio. I fornitori di servizi dei media audiovisivi e radiofonici, nel rispetto del principio di cui all'articolo 3 del citato regolamento e tenuto conto di quanto stabilito nel testo unico dei doveri del giornalista, osservano una serie di cautele e indirizzi, ponendo particolare attenzione all'identificazione del contesto specifico di riferimento rispetto a possibili rappresentazioni stereotipate e generalizzazioni, che, attraverso il ricorso a espressioni di odio, possono generare pregiudizio nei confronti di persone che vengano associate ad una determinata categoria o gruppo oggetto di discriminazione, offendendo così la dignità umana e generando una lesione dei diritti della persona. Il nuovo testo unico dei servizi dei media audiovisivi ha rafforzato i poteri dell'Autorità, introducendo, tra le disposizioni finalizzate a tutelare i diritti fondamentali della persona, l'articolo 30, a norma del quale i servizi dei media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi non devono contenere alcuna istigazione a commettere reati ovvero apologia degli stessi, in particolare: istigazione alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o di membri di un gruppo persone, sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o in violazione dell'articolo 604-*bis* del codice penale; alcuna pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo di cui all'articolo 5 della direttiva UE. Tanto premesso, spetta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigilare sull'eventuale presenza, nelle trasmissioni televisive trasmesse attraverso qualunque piattaforma, di contenuti lesivi della dignità umana e delle minoranze, che contengano incitamento all'odio basato sulla razza, sul sesso, sulla religione, sulla nazionalità, ed applicare, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi, in particolare quelli previsti dalle disposizioni in materia di tutela dei diritti fondamentali di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 208 del 2021, nonché dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana, secondo il quale tutti i cittadini hanno pari dignità sociale senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche. Per quanto concerne le iniziative di competenza dei Ministri interrogati, si evidenzia che il fenomeno del razzismo non deve essere sottovalutato; e in effetti non è sottovalutato. Al di là degli aspetti tecnici di questa risposta, che evidentemente non vogliono semplicemente delegare ad un'autorità terza il pronto intervento rispetto a comportamenti e linguaggi inadeguati, resta la coscienza della funzione che svolgiamo direttamente. Ciò vale per il Ministero che mi è stato affidato e vale naturalmente anche per il Ministero delle imprese e del Made in Italy. È sistematica la collaborazione con gli organismi competenti, perché possa essere più sviluppato il fattore di alfabetizzazione civico. È evidente che la principale alleata in questo tipo di impegno è, ancora una volta, la scuola, attraverso una collaborazione strutturata con il Ministero dell'istruzione e del merito, che rappresenta per noi in qualche maniera un punto di riferimento. non soltanto il razzismo, ma le discriminazioni in tutte le loro articolazioni devono essere anticipate con un'educazione che deve essere più puntuale. Resta inteso che l'educazione civica nella scuola, come stiamo effettivamente facendo, finalmente, dopo anni di abbandono culturale, debba essere il presidio principale, che vale per ogni tipo di comportamento inadeguato del ragazzo, dell'uomo e del cittadino in senso generale.

avvenuto nel corso di una partita di Lega Pro. Probabilmente la *gaffe* del telecronista, come ha riconosciuto il Ministro, è stata involontaria ed è stata colta da un pubblico anche assai ristretto. Tuttavia, anche in questa occasione, signor Ministro, come è ormai - ahimè - consuetudine, si è subito messa in moto la catena dei *social*, che si sono accaniti nei confronti del giovane centrocampista del Vicenza in ragione del colore della sua pelle. Questa è stata una cosa veramente grave e inaccettabile, proprio del risalto dato al mio atto di sindacato ispettivo, il telecronista si è affrettato a correre a Vicenza a stringere la mano e a scusarsi con Freddi Greco, quindi l'incidente è sicuramente chiuso, come egli ha riconosciuto, e va bene così. Tuttavia l'episodio ci fa capire come debba essere tenuta alta - e lei lo ha riconosciuto perfettamente - la guardia da parte del Governo, delle federazioni, degli agenti sportivi e di tutti coloro che hanno responsabilità nel mondo dello sport rispetto al fenomeno del razzismo, che anche in questo ambito deve essere punito con il massimo del rigore. Quello del razzismo non è certamente un fenomeno solo nostrano. Mi viene in mente, proprio recentissimamente, quanto denunciato qualche mese fa addirittura da un campione del Real Madrid, Vinícius, insultato nel campionato spagnolo. Bisogna lavorare a tutti i livelli affinché nessuno, da Vinícius a Freddi Greco, possa essere insultato in un campo da gioco per il colore della pelle. Ma le parole del Ministro ci rassicurano sull'impegno suo personale e dell'intero Governo su questo fronte. Mi consenta Ministro, forse extra politica ma da fruitore del mezzo televisivo: episodi anche recentissimi ci inducono a riflettere sulla professionalità, non sempre esemplare, delle nuove generazioni di telecronisti.

Signor Presidente, onorevoli senatori, rilevo in premessa che i termini riferiti usualmente alla carne, ai preparati o ai prodotti di carne (hamburger, bistecca, salame, eccetera) attualmente non godono, a livello nazionale ed europeo, di una specifica protezione o riserva, come invece previsto per quelli riferiti ai prodotti lattiero caseari. Riteniamo indispensabile, però, assicurare la corretta denominazione di tutti i prodotti che eviti qualsiasi confusione al cittadino e che garantisca la lealtà delle operazioni commerciali, in conformità all'articolo 7 del regolamento europeo n. 1169 del 2011. In particolare, le informazioni sugli elementi non devono indurre in errore circa la natura, l'identità, le proprietà, la composizione o evocare, tramite l'aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o ingrediente che, in realtà, è stato sostituito con un diverso componente o ingrediente. Al riguardo, ricordo che la Commissione europea, con comunicazione 2018/C 196/01 sull'applicazione dell'articolo 7 citato, ha precisato che: «Per quanto riguarda l'etichettatura di alimenti nei quali un ingrediente/ingredienti di sostituzione sono utilizzati all'interno di un prodotto, il nome del prodotto deve essere seguito nelle immediate vicinanze dalla denominazione dell'ingrediente/degli ingredienti di sostituzione, stampati sulla confezione o sull'etichetta in modo tale da garantirne la leggibilità e utilizzando un carattere la cui parte mediana (altezza della x) sia almeno pari al 75 per cento dell'altezza della x della denominazione del prodotto e che non sia inferiore a 1,2 mm». Per questa ragione sosteniamo tutte le iniziative parlamentari dirette a contrastare il fenomeno del *meat sounding*. Mi riferisco in particolare alla proposta di legge (Atto Camera 746) recante disposizioni in materia di denominazione dei prodotti alimentari contenenti proteine vegetali,

di alimenti e di mangimi sintetici, approvato in prima lettura al Senato il 19 luglio ultimo scorso. Il 25 luglio scorso il disegno di legge è stato assegnato all'esame delle Commissioni XII e XIII della Camera, assumendo la seguente rubrica: «Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali»,

al fine di salvaguardare e tutelare adeguatamente le produzioni nazionali che fanno della qualità una delle caratteristiche del *made in Italy*. In tale ambito, particolare attenzione viene riservata alle verifiche sull'etichettatura dei prodotti alimentari posti in commercio, tese a reprimere fenomeni di concorrenza sleali e assicurare al consumatore informazioni chiare e veritiere circa le caratteristiche dell'alimento, in particolare sulla natura, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il Paese di origine o il luogo di provenienza. Nel corso degli ultimi anni per prodotti vegetali o similari, l'Ispettorato ha eseguito 75 diffide per violazione delle disposizioni inerenti la presentazione dell'alimento ed elevato circa 20 contestazioni per violazione sulla denominazione e composizione di prodotti a base di carne o di prodotti lattiero-caseari, inclusi casi di non corretta etichettatura di prodotti presenti come analoghi al formaggio. Assicuro che l'Ispettorato continuerà a mantenere un elevato livello di attenzione sui prodotti posti in commercio, sia sul mercato reale nazionale che nei siti di vendita *online*, al fine di garantire la veridicità delle informazioni fornite al cittadino, di evitare fenomeni distorsivi del mercato e di concorrenza sleale per quanto riguarda il settore delle carni.

Facciamo un breve ragionamento e iniziamo a dire che c'è un'enorme differenza tra i prodotti a base vegetale e i prodotti sintetici, quelli prodotti in laboratorio di cui abbiamo parlato parlato anche in queste Aule. I prodotti a base vegetale sono prodotti naturali, che servono a dare una risposta a tutta quella fascia di popolazione, molto ampia nel nostro Paese, che

relativa - come abbiamo sempre detto - ai prodotti di laboratorio, sui quali non c'è ancora una specifica indicazione, neanche da parte del mondo sanitario, che ci dica esattamente se fanno bene o fanno male, nonostante alcune rassicurazioni che abbiamo ascoltato durante le audizioni alla Camera dei deputati, ma sono

lunghissimo di prodotti che possono portare il consumatore in errore: hamburger di ceci e zucchine, hamburger vegano, hamburger di lenticchie, hamburger di fagioli, hamburger di spinaci e hamburger di melanzane, polpette di ceci, polpette di verdura, wurstel vegetariani, hot-dog vegano, cotoletta vegana, salame vegano, salsiccia di ceci, bresaola vegan, bistecche di qualsiasi tipo. Potrei veramente andare avanti, ma non mi metto a parlare di latte e di prodotti da esso derivati. In questo momento c'è veramente la necessità di fare estrema

Penso che siamo sulla buona strada per tutelare i consumatori, soprattutto, ma anche i produttori che, in questo momento, con il *meat sounding* che si aggiunge all'*italian sounding* e a tutto quello che sta un po' devastando il nostro agroalimentare, hanno bisogno di essere *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*.

Signor Presidente, ringrazio gli onorevoli interrogati per il tema sollevato che mi consente di chiarire alcuni aspetti riguardanti le azioni intraprese a favore dei lavoratori del settore della vigilanza privata. I servizi ausiliari della sicurezza erogati da risorse qualificate sono essenziali per garantire la salvaguardia e l'efficienza di un patrimonio sia materiale che immateriale. Nel settore della vigilanza dei servizi fiduciari le retribuzioni del personale impiegato nei servizi risultano tuttavia estremamente basse. Il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro costituisce una prerogativa delle parti sociali che nell'esercizio della loro autonomia negoziale stipulano e rinnovano con la necessaria regolarità gli strumenti di contrattazione collettiva. Consapevoli che la contrattazione collettiva deve essere rinforzata e valorizzata, di recente abbiamo proceduto alla convocazione di uno specifico tavolo per esaminare le problematiche del settore con particolare riguardo ai salari del personale non armato, *in primis* la committenza pubblica che rappresenta una quota consistente degli appalti di servizi in corso è chiamata con forza a svolgere la sua parte nell'ottica di un progressivo e concertato innalzamento dei livelli retributivi. A tal fine, già dai prossimi giorni, riprenderà un ciclo di incontri con le parti sociali che possa consentire un continuo e progressivo adeguamento dei livelli salariali previsti nella contrattazione collettiva nazionale di settore rinnovato il 6 luglio ultimo scorso. La particolare condizione economica nonché l'insostenibilità di molte offerte economiche degli appalti di servizi ad alta intensità di lavoro umano deve condurre una serie di azioni volte a sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori nel settore della vigilanza e dei servizi fiduciari e la sostenibilità dei costi per le imprese del settore. Infine per quanto riguarda l'estensione della legge n. 66 del 2023 nel settore della vigilanza, il Ministero manifesta la disponibilità ad approfondire le questioni con gli uffici tecnici competenti, atteso che la disciplina di organizzazione dell'orario di lavoro, regime dei riposi, ferie, eccetera,

portato a qualcosa più di 6 euro. Si sta cercando di capire come poter riavvicinare questo loro rinnovo. Siamo convinti che le stesse pubbliche amministrazioni che in qualche modo costruiscono la gara d'appalto non si possano permettere di pagare così poco questo personale. Lavoreremo allora per far sì che anche nella pubblica amministrazione le gare d'appalto non vengano fatte con queste tabelle.

Grazie,

Successivamente alla sigla del contratto di giugno, come avete letto sui giornali, sono state commissariate tre importanti aziende del settore: mi riferisco alla cooperativa Sicuritalia, a Mondialpol, a Cosmopol,

alla scadenza del contratto previsto ad aprile 2026. Siamo quindi sicuramente a livelli inferiori rispetto al salario minimo proposto di 9 euro, che è già in vigore in tanti contratti collettivi nazionali. So che il sottosegretario Durigon oggi incontrerà i sindacati in un tavolo, quindi le chiedo direttamente di farsi portavoce di rivedere il contratto nazionale collettivo appena siglato e di farsi direttamente promotore di un nuovo contratto collettivo sulla base di quanto diceva, anche per la decenza di questi dipendenti, per prevedere un contratto collettivo, anche magari copiandolo

una nuova finestra"). L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.

*(M5S)*. Signor Ministro, finalmente, dopo tanti annunci da parte sua e da parte della *Premier*, la sera del 19 settembre è stato pubblicato in Gazzetta il decreto in cui si scrive nero su bianco che intendete procedere con il progetto di realizzazione di tanti centri per il rimpatrio (CPR) su tutto il territorio nazionale, tanto da averne uno per per ogni Regione. La pubblicazione di questo decreto, piuttosto che diradare le nebbie, purtroppo le ha infittite, perché infatti non si capisce per per chi si vogliono costruire questi CPR, dato che nel decreto Cutro, annunciato in pompa magna nello stesso luogo di quella terribile tragedia per la quale ancora si cercano le responsabilità - a questo proposito, Ministro, le chiedo anche, per favore, di riferire quanti trafficanti avete acciuffato alla fine, dopo averli inseguiti in tutto il globo terracqueo - avete stabilito che nei CPR ci possono finire anche i richiedenti asilo. In altre sedi, invece, dite che nei CPR ci possono finire soltanto i destinatari di decreto di espulsione. le chiedo di chiarire agli italiani, per favore, per chi volete trasformare l'Italia in un enorme *hotspot* di carceri a cielo aperto. Ma c'è di più: anche l'aspetto dei costi non è chiaro, perché nel decreto si parla di 20 milioni, di 20 milioni, ma avendo voi innalzato anche il termine di trattenimento fino ad un massimo di diciotto mesi, oggi in Italia abbiamo nove CPR per 619 posti disponibili; aumentandoli di 12 si può arrivare a circa 2.000 posti. Ma i rimpatri, come lei sa, si possono effettuare soltanto attraverso accordi bilaterali che l'Italia purtroppo praticamente non ha, per cui su 28.000 decreti di espulsione del 2022 ci sono stati soltanto pertanto, quanto costerà questo progetto che prevede la costruzione di tutti questi centri e il loro mantenimento a lungo termine sia in termini economici, gestionali, e quale risultato concreto sperate di raggiungere considerata l'assenza degli accordi bilaterali di cui sopra.

Signor Presidente, con il decreto-legge che è stato richiamato dall'onorevole interrogante è stato esteso il periodo di permanenza degli stranieri nei centri per il rimpatrio introdotti - lo voglio ricordare - dalla legge cosiddetta Turco-Napolitano fino ad un massimo di diciotto nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento sia durata più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte dello straniero o a causa dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dei Paesi terzi. Si tratta di un intervento coerente con il vigente quadro normativo dell'Unione europea, che prevede la possibilità del trattenimento fino a diciotto mesi degli stranieri destinatari dell'espulsione dal territorio nazionale. Relativamente al trattenimento dei richiedenti asilo nei CPR, preciso che si tratta di una eventualità che è già prevista dal decreto legislativo n. 142 del 2015 di recepimento di direttive europee, in relazione a casi riconducibili ad esigenze primarie di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. Ciò premesso, è opportuno sottolineare che il 70 per cento dei soggetti rimpatriati ad oggi è transitato per un CPR. Ad oggi, circa il 50 per cento degli stranieri che vi vengono trattenuti viene rimpatriato. Questi dati indicano una forte correlazione tra il numero dei rimpatri e i posti disponibili nei CPR, che oggi sono insufficienti. Tale evidenza è alla base della decisione di realizzare nuovi CPR sul territorio nazionale e di ripristinare la piena funzionalità delle strutture esistenti. è aprire almeno un centro in ogni Regione e, a tal fine, il recente decreto-legge n. 124 prevede un piano straordinario per l'individuazione delle aree interessate alla realizzazione di un numero idoneo di strutture anche attraverso la valorizzazione di immobili già esistenti. L'inserimento dei CPR in tale piano ci consentirà di avvalerci delle procedure speditive e in deroga già previste per le opere destinate alla difesa nazionale, e a questo scopo sono stati stanziati 20 milioni di euro - lo ricordava lei - per l'anno in corso; ma il piano potrà essere aggiornato periodicamente anche sotto il profilo delle risorse necessarie. Inoltre, al fine di rendere effettivi i rimpatri di coloro che non hanno titolo a permanere sul territorio nazionale, stiamo lavorando sul piano della collaborazione internazionale per incrementare gli accordi con i Paesi di origine e contemporaneamente per comprimere i tempi del procedimento di espulsione. Circa i dati relativi all'attività di contrasto, dall'entrata in vigore del cosiddetto decreto-legge Cutro il totale degli arresti per favoreggiamento dell'immigrazione irregolare ammonta a cento persone; il totale delle imbarcazioni sequestrate per favoreggiamento dell'immigrazione irregolare è di 368; gli arresti fatti dalla sola Guardia di finanza per il reato di pirateria sono ben dieci, e nella contestazione di questo reato ben due imbarcazioni sono state sequestrate dalla Guardia di finanza. Voglio chiudere ringraziando le forze dello Stato, la Guardia di finanza, la Marina militare, le Capitanerie di porto, che stanno conciliando, con la loro incessante attività, la salvaguardia della vita delle persone con un'importante azione di contrasto e di deterrenza in uno scenario operativo particolarmente difficile.

verranno costruiti - sono nulla rispetto ai 132.000 sbarchi che, ad oggi, si registrano a seguito del grandissimo successo del decreto vergogna

davvero questo provvedimento nasce già pasticciato, al punto da aver sollevato un dibattito incredibile anche con i vostri stessi Presidenti di Regione: alzare il telefono e chiamare i vostri stessi Presidenti di Regione, con Zaia che dice «io non ne so niente e comunque pavento criticità sociali», Giani che ha già detto «no, grazie», altri che hanno detto sì, e lei che dice «dialogheremo con tutti ma imporremo la nostra linea», senza neanche rendersi conto del controsenso di quanto afferma. Signor Ministro, la prego: basta propaganda, vi siete resi conto che occorre diplomazia in Europa e nei Paesi di origine. Speriamo davvero che questo si sia capito.

- Premesso che: le stazioni ferroviarie e le relative aree limitrofe si trasformano troppo spesso in luoghi pericolosi e degradati, dove si sviluppano fenomeni di emarginazione, di delinquenza e di violenza e dove la percezione di insicurezza è molto diffusa; in questi giorni sono stati siglati accordi in diverse città italiane per la promozione della sicurezza integrata nelle stazioni ferroviarie con lo scopo di assicurare, in particolare nelle ore notturne, specifici servizi all'interno degli scali, quando essi non sono presidiati dalla Polizia ferroviaria; negli ultimi mesi sono state intensificate le attività di prevenzione, controllo e contrasto alla microcriminalità nelle zone adiacenti alle stazioni ferroviarie, a partire da Roma, Milano e Napoli, con l'obiettivo di assicurare una presenza rafforzata e visibile delle forze di polizia e offrire una più efficace risposta al bisogno dei cittadini di protezione;

degrado ed emarginazione e, conseguentemente, criminalità e violenza; è assolutamente necessario mettere in atto azioni concrete nelle aree a più alto rischio criminalità, che siano quelle adiacenti agli scali ferroviari o quelle periferiche con condizioni di degrado e marginalità sociale in cui le organizzazioni criminali trovano terreno fertile soprattutto tra i giovani, sicuramente attraverso il presidio della sicurezza e della legalità, ma anche con risposte sul piano sociale, educativo, culturale, delle infrastrutture sportive, che offrano opportunità e alternative ai ragazzi; si assiste con troppa frequenza su tutto il territorio nazionale ad aggressioni violente e immotivate da parte di ragazzi, anche giovanissimi: il fenomeno delle *baby gang* rappresenta oggi una vera e propria emergenza sociale, che deve essere gestita congiuntamente dalle diverse istituzioni coinvolte, di sapere quali siano i risultati degli interventi di prevenzione, controllo e contrasto alla criminalità messi in atto negli ultimi mesi per garantire la sicurezza nelle aree periferiche delle città italiane, in particolare nelle zone limitrofe alle stazioni ferroviarie, e quali siano le azioni programmate per proseguire, ampliare e potenziare tali interventi, anche prevedendo

Signor Presidente, fin dal mio insediamento ho dedicato una particolare attenzione, com'è noto, alla sicurezza nelle città, attivando un *forum* con i sindaci delle città metropolitane proprio sui temi della sicurezza urbana e presiedendo personalmente molteplici Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica. In questa direzione si inquadrano le operazioni ad alto impatto che stanno aumentando le nostre capacità di controllo dei luoghi pubblici ad elevata concentrazione di persone, come le stazioni, le aree urbane della cosiddetta movida e le piazze di spaccio. Anche la mia direttiva ai prefetti dopo i fatti di Caivano si inserisce in questo percorso, essendo rivolta ad acquisire un'aggiornata ricognizione sull'intero territorio nazionale delle aree caratterizzate dalle più gravi forme di degrado, sulle quali intervenire con analoghe misure, garantendo una presenza visibile e rafforzata dello Stato e delle Forze di polizia. Cito i dati. A partire dall'inizio dell'anno, nelle sole città di Roma, Milano, Napoli, Torino, Firenze, Bologna, Bari e Palermo, sono state impiegate circa 40.000 unità delle forze di polizia, che hanno potuto contare sul supporto di oltre 5.000 unità di polizia locale, operatori delle aziende sanitarie locali, aziende municipalizzate ed ispettorati del lavoro. Sono state effettuate 633 operazioni ad alto impatto; di queste, 288 sono state svolte nelle stazioni ferroviarie e nelle aree limitrofe delle città coinvolte e 345 in zone urbane degradate. Sono state controllate più di 359.000 persone, di cui 766 arrestate e 4.524 denunziate. Sono stati adottati quasi 900 provvedimenti di espulsione nei confronti di cittadini stranieri, controllati oltre 44.000 veicoli e circa 8.300 esercizi pubblici. D'intesa con i Ministri della difesa e delle infrastrutture e trasporti stiamo mettendo appunto un piano di intervento dei militari a supporto delle Forze di polizia impegnate negli specifici servizi di controllo delle stazioni ferroviarie delle principali città, con una integrazione significativa del contingente delle Forze armate delle operazioni strade sicure. Per quanto poi riguarda le cosiddette *baby gang*, con il recente decreto-legge 123, all'esame di questo ramo del Parlamento, sono state introdotte misure per il contrasto alla violenza minorile, quali l'estensione del daspo urbano, l'affinamento dell'avviso orale del questore, nonché pene più severe per i reati in materia di armi e stupefacenti, ma anche misure volte a rafforzare l'offerta scolastica e a combattere l'abbandono precoce della scuola, quale parte integrante di un'azione sistematica di prevenzione del disagio giovanile. La strategia del Governo, recependo anche le indicazioni emerse in sede dei Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica presso le Prefetture, che vengono allargati alla partecipazione di tutte le componenti istituzionali interessate, si sta muovendo su più piani, con azioni di breve, medio e lungo periodo, che affiancano alle operazioni di contrasto iniziative sul piano economico, sociale, educativo e culturale, volte a riqualificare le nostre città e ad affermare pienamente... Non si tollerano zone franche nel nostro Paese. per ripristinare la legalità, la sicurezza e anche il decoro nelle nostre stazioni e nelle zone adiacenti, per la sicurezza dei milioni di cittadini italiani che usano il treno tutti i giorni, ma anche per i milioni di turisti che arrivano nel Paese più bello del mondo e che si sono trovati per anni davanti a degli scenari orribili e inaccettabili di insicurezza e di degrado: tossicodipendenti, ubriaconi che litigano tra di loro, tassisti abusivi, senzatetto che urinano indisturbati davanti a tutti, ladri e spacciatori. Anche chi chiede l'elemosina lo stava iniziando a fare in modo sempre meno garbato e sempre più pretenzioso e fastidioso, obbligando i passeggeri, anche quelli in fila per i taxi, a fare lo zig-zag tra questi. Il piano fatto ad inizio anno, d'intesa tra lei e il ministro Salvini, che prevede l'assunzione di persone nei prossimi anni destinate alla sicurezza delle stazioni, gli investimenti per i tornelli e per i *gate*, le misure che lei ha annunciato oggi qui e che ha già messo in campo negli ultimi mesi consentiranno di porre riparo e rimedio a una politica buonista follemente cieca, più che tollerante, del centrosinistra, che ancora amministra le tre grandi città italiane, con risultati che sono sotto gli occhi di tutti.

Signor Ministro, nell'ultimo anno gli sbarchi sull'isola di Lampedusa sono aumentati e la situazione è diventata vieppiù critica. L'*hotspot* versa in condizioni inaccettabili di grave sovraffollamento e di estremo degrado. I sindaci e le amministrazioni locali sono stati lasciati soli, senza risorse e senza strumenti normativi adeguati. Il numero delle persone giuridicamente irregolari presenti in Italia è aumentato. In Europa, i Governi con i quali condividete le pulsioni sovraniste e nazionaliste più radicali, come ad esempio il Governo polacco e quello ungherese, hanno ostacolato e stanno ostacolando qualsiasi risposta europea condivisa, a partire da una riforma del regolamento di Dublino o dall'adozione di una Mare Nostrum europea. I naufragi e le morti intanto proseguono. Ecco, signor Ministro, noi vorremmo sapere innanzitutto se sono questi gli obiettivi che intendevate conseguire con la retorica e la demagogia della sovranità, del "prima gli italiani", e con l'adozione dei decreti n. 1 e n. 20 del 2023, 2023, con i quali - lo voglio ricordare - avete prima preso di mira le ONG, obbligandole ad esempio a recarsi, senza ritardo, in porti anche molto lontani dall'area in cui è avvenuta l'operazione di soccorso e a non effettuare quindi salvataggi multipli. Poi, con il decreto Cutro, avete disposto un'incomprensibile restrizione della protezione speciale, avete ridotto le garanzie giurisdizionali e avete ipotizzato di moltiplicare i CPR e di allungare i tempi di trattenimento, senza naturalmente prestare alcuna attenzione alle condizioni in cui sono costrette le persone in tali centri. Ma, oltre a questa domanda, tutt'altro che retorica, signor Ministro, e drammaticamente seria, le chiediamo di sapere in particolare quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di contrastare in modo efficace il traffico di esseri umani, prevedendo nuovi canali di ingresso legale in tutti i Paesi dell'Unione europea, sia per coloro che chiedono protezione internazionale, sia per coloro che sono in cerca di lavoro, poiché le vie legali e sicure per l'ingresso rappresentano l'unica alternativa efficace al traffico di esseri umani. Poi le chiediamo di sapere quali iniziative intenda adottare, di concerto con i sindaci e le amministrazioni comunali, per realizzare un piano efficace di accoglienza diffusa. E, ancora, come intenda dare piena ed effettiva attuazione alla legge n. 17 del 2017, la cosiddetta legge Zampa, in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Ecco, noi vorremmo, signor Ministro, che lei desse a noi e al Paese una risposta seria.

in modo esauriente sarebbe stato necessario un tempo assai più ampio di quello a mia disposizione, però farò del mio meglio, evidenziando in primo luogo che l'impennata dei flussi di questi ultimi mesi non ci ha affatto colto impreparati. La dichiarazione dello stato di emergenza dello scorso aprile e ancor prima le misure contenute nel decreto-legge n. 20 del 2023, ci hanno consentito di programmare per tempo il miglioramento della nostra capacità di risposta ad una situazione di eccezionale complessità. Abbiamo completamente riorganizzato la gestione dell'*hotspot* di Lampedusa e di altri *hotspot* in Sicilia e Calabria, per assicurare la continuità e la rapidità dei massicci trasferimenti dei migranti giunti via mare, alleggerendo la pressione soprattutto su Lampedusa, ove per garantire i migliori servizi di accoglienza, la gestione dell'*hotspot* è stata affidata alla Croce Rossa Italiana. Contemporaneamente, in pochi mesi abbiamo aumentato del 10 per cento i posti in accoglienza ed implementato la rete degli *hotspot* in Sicilia ed in Calabria, con oltre 3.000 nuovi posti, così da attenuare l'impatto dei massicci afflussi sul restante territorio nazionale. Attualmente il sistema di accoglienza nazionale ospita oltre 136.000 persone di cui circa 35.000 nella rete SAI, oltre 95.000 nei CAS per adulti, quasi 1.400 nei CAS per minori e circa 4.800 nei centri di prima accoglienza. Le persone in accoglienza sono distribuite in 6.114 strutture CAS adulti e minori e in 926 progetti SAI con il coinvolgimento complessivo di quasi 3.000 Comuni. Si tratta di dati che dimostrano chiaramente il livello di capillarità dell'accoglienza su tutto il territorio nazionale, con evidenti benefici anche sull'ordine pubblico. Nel loro insieme, le misure intraprese dal Governo in materia migratoria stanno colmando un *deficit* di pianificazione che si è protratto negli anni e stanno permettendo di adeguare rapidamente il sistema di accoglienza alle esigenze della eccezionale pressione migratoria. Oltre a ciò, è stato dato nuovo impulso ai corridoi umanitari - oltre mille rifugiati accolti, più di qualsiasi anno precedente - e all'immigrazione legale dei lavoratori stranieri attraverso l'ampliamento delle quote di ingresso, portandole ad oltre 136.000 per l'anno in corso. E abbiamo anche introdotto una programmazione triennale delle quote per meglio corrispondere alle esigenze del mercato del lavoro e favorire iniziative di collaborazione più a lungo termine con i Paesi d'origine dei flussi, arrivando ad un totale di 452.000 unità. Anche questo non è stato fatto negli anni precedenti. Quanto alle iniziative sul piano internazionale, l'Italia si sta adoperando su tutti i tavoli negoziali al fine di ottenere una efficace gestione europea dei flussi migratori e nuove regole basate su maggiore equilibrio tra responsabilità dei Paesi di primo ingresso e solidarietà degli Stati membri. Proprio nella direzione di rivedere anche i rigidi criteri del cosiddetto regolamento di Dublino vanno i risultati sinora ottenuti nel Consiglio giustizia e affari interni dello scorso 8 giugno, tra i quali proprio la mitigazione del principio di responsabilità esclusiva dello Stato di primo ingresso e la creazione di un nuovo Fondo europeo a favore dei Paesi di origine e transito dei flussi, risultati riconducibili ad una precisa spinta negoziale impressa proprio dall'attuale Governo.

collegati ad una politica complessiva della migrazione che noi non vediamo. Anzi, il fatto di continuare ad avere delle risposte frammentate su singoli aspetti è uno dei problemi che osserviamo. Nella sua risposta, lei ha dato dei numeri ha detto che il sistema dell'accoglienza funziona e che addirittura ci sono benefici sull'ordine pubblico. Allora viene da chiedersi perché, proprio nel momento in cui ci sono i risultati positivi da lei asseriti, anche anche sull'ordine pubblico, si prevede di moltiplicare i CPR. È una contraddizione che lega ancora la questione della migrazione, confondendo soccorso, accoglienza, integrazione, respingimenti ed espulsioni. Lei non ha risposto sulla ipotesi di un Mare nostrum, non ha risposto sulla domanda relativa

che vi è il diritto a restare in un Paese anche da parte di coloro che vi si trovano, non avendo ancora valicato una frontiera. Sono questioni generali, complesse, difficili ma la risposta che ci sembra diate è quella di continui decreti. Il fatto di continuare a produrre decreti su decreti in qualche misura evidenzia che la politica che intraprende questo Governo è forse legata più agli appuntamenti elettorali che non ad una vera volontà di affrontare il tema del suo complesso. Noi abbiamo posto un'altra domanda importante che riguarda che cosa farà lei a proposito della cosiddetta legge Zampa, dei moltissimi minori che hanno il diritto di restare e di poter essere trattati diversamente anche coinvolgendo i Comuni e tutte le associazioni locali. Mi sono recato qualche giorno fa a Rosolini, in un centro

tutte le questioni complessivamente, dal soccorso all'accoglienza; ci meraviglia che ci sia questa pressione su Lampedusa e che non ci sia uno smistamento organizzato in tutte in tutte le altre fonti di accoglienza nazionali, considerato quanto lontano vengono mandate poi le navi delle ONG. Noi riteniamo che questa politica fatta di decreti successivi sia sbagliata e contraria al rispetto della dignità delle persone, a questo punto non soltanto di quelle soccorse, ma anche di coloro che rappresentano chi li soccorre.

signor Ministro, colleghi, sottopongo oggi all'attenzione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica una questione di grande interesse per gli italiani. Parliamo di energia e di mercato tutelato. Ad oggi gli utenti di luce e gas si dividono tra coloro che sono già passati al mercato libero dell'energia, aderendo a una delle offerte pubblicizzate dai vari fornitori, e coloro - circa 10 milioni di clienti domestici - che sono rimasti nel cosiddetto mercato tutelato, godendo cioè di condizioni economiche definite dall'Authority dell'energia. Il 10 gennaio 2024 finisce il mercato tutelato dell'energia; chi è già passato o passerà nei prossimi mesi al mercato libero non sarà chiaramente interessato da alcun cambiamento, ad eccezione dei clienti vulnerabili ovvero delle persone con disabilità, di chi si trova in condizioni di salute tali che richiedono l'utilizzo di apparecchiature medico terapeutico salvavita, chi si trova in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi e di chi abita chiaramente in un'isola minore non interconnessa. Tutti gli altri - come dicevo prima, circa 10 milioni di italiani - finiranno nel cosiddetto servizio a tutele graduali. Di cosa si tratta? Il fornitore sarà selezionato dall'ARERA tramite un'asta, l'Italia sarà suddivisa in 26 zone e per ogni zona ci sarà un vincitore di tale asta. Sarà un regime transitorio che durerà tre anni, da aprile 2024 ad aprile 2027, al termine del quale sarà obbligatorio il passaggio al mercato libero. Si tratta di un cambiamento importante che va gestito con la massima attenzione perché ogni offerta del mercato libero è più o meno vantaggiosa per un utente in base ai suoi consumi e alle sue abitudini di utilizzo. Ecco dunque che diventa importante - è questa la richiesta che oggi rivolgo rivolgo al Governo e a lei signor Ministro - informare - ribadisco informare - i cittadini. Il nostro obiettivo è e rimane tutelare le famiglie, soprattutto quelle meno abbienti. Non a caso, infatti, il Governo nel 2022 ha speso 40 miliardi di euro per contenere l'aggravio dei costi dell'energia per famiglie e imprese. Sono circa 7 milioni e mezzo le famiglie in difficoltà economica che hanno beneficiato finora dei *bonus* sociali. Tornando al tema al centro dell'atto di sindacato ispettivo di oggi in esame, il passaggio verso il mercato libero dell'energia dal 2027 pone delle questioni che vanno certamente affrontate. Si rende necessario garantire le famiglie italiane rispetto alla fine del mercato tutelato. Chiediamo quindi a lei, signor Ministro, di sapere quali siano le azioni che il Governo intende intraprendere per assicurare un'adeguata informazione a sostegno della fine del mercato tutelato ai clienti domestici.

è in fase di attuazione l'ultimo *step* della cessazione del regime di maggior tutela che coinvolge i cosiddetti clienti domestici. Il Governo è conscio della rilevanza di questo passaggio e in particolare dell'importanza di accompagnare tale cambiamento con un'adeguata attività di informazione, affinché si promuova la massima consapevolezza da parte degli utenti e il completamento della liberalizzazione del mercato rappresenti un reale beneficio per gli stessi. Sulla base dei principi fissati dalla decretazione ministeriale, saranno svolte campagne di comunicazione istituzionale su larga scala attraverso una pluralità di canali divulgativi e sui principali *media* a diffusione nazionale, reti e ambiente (ARERA) e con il supporto dell'acquirente unico. Ciò al fine di veicolare le corrette informazioni sulla normativa vigente in materia di apertura del mercato, sulle caratteristiche del servizio a tutele graduali, sulle relative tempistiche, sugli obblighi e sui diritti dei clienti finali, nonché sulle opportunità del mercato in termini di potenziali vantaggi derivanti da una pluralità di offerte trasparenti e confrontabili. Gli utenti dovranno essere informati degli strumenti a loro disposizione per una scelta consapevole dei fornitori, delle offerte e degli strumenti di tutela. Le azioni saranno messe in campo nei tempi utili e necessari a garantire la piena efficacia degli interventi (quindi con adeguato anticipo), nonché in prossimità dell'effettivo trasferimento dei punti di fornitura ai nuovi esercenti assegnatari del servizio a tutele graduali, in modo da sollecitare efficacemente la scelta attiva da parte del cliente. È inoltre previsto che gli utenti ricevano opportune comunicazioni per il tramite della bolletta elettrica sulla base di quanto sarà stabilito dall'autorità di regolazione, chiamata altresì a rafforzare la trasparenza e la chiarezza informativa sulle condizioni di fornitura e sui prezzi, in modo da agevolare il confronto autonomo dei clienti tra le offerte economiche di tutela e le alternative disponibili sul mercato. Sono in corso valutazioni da parte del Governo sul meccanismo di traghettamento al di fuori del mercato tutelato dei clienti domestici e in particolar modo dei vulnerabili, tenendo conto dell'instabilità dei prezzi dell'energia in questa fase storica. Si stanno valutando tempi e modalità del trasferimento.

dal mercato tutelato a quello libero è certamente indispensabile - come diceva il signor Ministro - mettere in atto una capillare ed efficace campagna di comunicazione su larga scala sui principali *media* nazionali attraverso una pluralità di canali, con l'obiettivo di promuovere una scelta consapevole dei fornitori di luce e gas da parte delle famiglie stesse. Le parole del Ministro ci confermano l'attenzione di questo Governo e di questa maggioranza nei confronti delle famiglie proprio sulla questione del caro energia. Come giustamente evidenziato, c'è bisogno di trasparenza e chiarezza informativa per promuovere una scelta consapevole da parte di tutti i cittadini. Al tempo stesso auspichiamo, vista l'instabilità dei prezzi dell'energia in questa fase storica, il massimo impegno sulle famiglie meno abbienti, con le misure di sostegno adeguate e necessarie.

Signor Ministro, lei sa bene che ci troviamo in una fase particolare del contesto storico in cui si intrecciano diverse crisi (quella climatica, quella energetica e quella internazionale) e c'è un evidente collegamento tra i temi tra i temi dell'approvvigionamento energetico e della giustizia climatica e il tema della sicurezza internazionale. La guerra in Ucraina ci ammonisce di quanto l'Italia e l'Europa debbano non solo diversificare le fonti di produzione dell'energia, ma anche garantire la produzione *in loco*, nel nostro territorio, così da essere meno esposte a un uso geopolitico delle risorse le comunità energetiche e l'autoconsumo collettivo pongono le basi per una distribuzione diffusa e generata dell'energia, in cui la produzione delle fonti rinnovabili *in loco* consente di ridurre il rischio di dipendenza dai combustibili fossili. Il GSE il 15 giugno del 2023 ha accolto 74 richieste per 21 CER (Comunità energetiche rinnovabili) e 53 gruppi per l'autoconsumo collettivo. Le 21 CER includono 28 impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di circa 430 chilowattora e coinvolgono complessivamente 163 punti di prelievo prevalentemente nella titolarità di persone fisiche, piccole e medie imprese e Comuni presenti in appena sei CER. I 53 gruppi per l'autoconsumo collettivo includono 67 impianti per una potenza complessiva di circa 1,1 megawatt, nonché 381 punti di prelievo.

le chiedo a che punto siamo rispetto all'attuazione di questo decreto dal quale dipende la Comunità energetica rinnovabile di molti territori: penso alla Lombardia, con la quale lavoriamo insieme alla collega, senatrice Gelmini; penso alla Toscana, all'Emilia-Romagna, alla Calabria e a tutte le Comunità energetiche che aspettano

siamo nella fase finale delle interlocuzioni con la Commissione europea nell'ambito dell'*iter* di valutazione della compatibilità della misura proposta con la normativa in materia di aiuti di Stato. Le interlocuzioni con la Commissione sono state costanti e proficue sin dalla necessaria fase di pre-notifica (dal 15 marzo) avviata addirittura lo scorso febbraio e dettata dalla particolare complessità dello schema di decreto - che è una novazione anche a livello europeo che disciplina, sia la concessione di una tariffa incentivante a valere sull'energia elettrica prodotta e condivisa all'interno delle configurazioni di autoconsumo, sia la concessione di ingenti contributi di PNRR in conto capitale nell'ambito dei Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti. La misura in argomento prevede, inoltre, l'accesso al meccanismo di supporto diretto senza la necessità di richiedere la preventiva iscrizione a bandi o registri. Peraltro, lo scorso 28 luglio la Commissione ha formulato una formale e approfondita richiesta di informazioni che ha avuto riscontro in data 11 settembre e vi è stata altresì una discussione in dettaglio con gli uffici della Commissione *de visu*

alla parte impresa - e predisporre le opportune revisioni del testo, che sono state già definite, che, una volta avallate dalla Commissione europea, permetteranno di attivare questa rilevante misura nel percorso di decarbonizzazione del nostro Paese.

che non c'è nessun profilo di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea, in particolare con il tema degli aiuti di Stato, ma non posso essere soddisfatto dall'affermazione che siamo nella fase finale, perché, come lei sa bene e come emerge anche dalla sua risposta, le comunità energetiche rinnovabili hanno bisogno di un termine preciso entro il quale dare la decretazione che consenta loro di stimolare la produzione energetica *in loco* e quindi ci potremo definire soddisfatti come Gruppo solo quando al riferimento alla fase finale dell'interlocuzione

signor Ministro, colleghi, il dibattito intorno alla necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento energetico, scatenato in particolare dal conflitto russo-ucraino e dal conseguente forte rialzo dei prezzi del gas, ha riportato l'attenzione anche sul tema dell'energia nucleare, il tema dell'energia nucleare è di recente tornato d'attualità anche in seguito a quanto proposto dalla Commissione europea, di inserire tale forma di produzione di energia nella tassonomia degli investimenti sostenibili, è fondamentale valutare tutte le soluzioni possibili per accelerare la transizione energetica e raggiungere gli obiettivi climatici al 2030 e al 2050;

la "piattaforma" costituirà il soggetto di raccordo e coordinamento tra tutti i diversi attori nazionali che a vario titolo si occupano di energia nucleare, sicurezza e radioprotezione, rifiuti radioattivi, sotto tutti i profili. In particolare, si punta allo sviluppo di tecnologie a basso impatto ambientale e ad elevati *standard* di sicurezza e sostenibilità,

che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso alla Commissione europea già indica che le tecnologie nucleari di nuova generazione svolgeranno un ruolo importante nella transizione energetica verso un'economia a bassa emissione di gas serra. Pertanto, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione assunti dal nostro Paese e con la mozione approvata lo scorso maggio dal Parlamento italiano, il Ministero ha istituito la Piattaforma nazionale per un nucleare sostenibile. Questa mattina presso il Ministero si è svolta la prima riunione della Piattaforma. L'incontro ha visto la partecipazione dei principali enti pubblici di ricerca, di esponenti rappresentanti il mondo dell'università, di associazioni scientifiche, di soggetti pubblici operanti nel settore della sicurezza nucleare, del *decommissioning*, nonché di imprese che hanno già in essere programmi di investimento nel settore nucleare, nella produzione di componenti e impianti e nelle applicazioni mediche nel settore nucleare. e di Ricerca per il sistema energetico (RSE), si pone l'obiettivo di definire in tempi certi un percorso finalizzato alla possibile ripresa dell'utilizzo dell'energia nucleare in Italia e alle opportunità di crescita della filiera industriale nazionale già operante nel settore. L'obiettivo prioritario sarà quello di sviluppare nell'arco di alcuni mesi delle linee guida e una *road map* con l'orizzonte del 2030 e del 2050 per seguire e coordinare gli sviluppi delle nuove tecnologie nucleari nel medio e nel lungo termine, con particolare attenzione agli *small modular reactor* e ai reattori di quarta generazione, nonché comprendere le possibili ricadute di queste tecnologie in termini di sicurezza e rapporto costi-benefici del sistema. Infine, in relazione alla tecnologia della fusione, occorrerà valutare nel lungo termine il supporto che sarà in grado di dare alle energie rinnovabili per il raggiungimento dei *target* previsti nell'aggiornamento del Piano I risultati del lavoro della piattaforma saranno la base per valutare l'elaborazione e l'adozione da parte dell'Italia di una strategia nazionale per il nucleare sostenibile.

che, in particolare, l'ENI vuole puntare molto sulla fusione nucleare perché, come ha detto l'amministratore delegato Descalzi, permette di ottenere energia pulita, inesauribile e sicura per tutti: una vera rivoluzione, capace di superare le diseguaglianze fra le Nazioni e di favorire la pace. Descalzi ha poi aggiunto che nel 2025 2025 sarà pronto un impianto pilota a confinamento magnetico in grado di ottenere elettricità dalla fusione e che nel 2030 sarà operativa la prima centrale industriale basata su questa tecnologia. Non possiamo che rallegrarci per obiettivi così ambiziosi. Credo però che il Governo anche per il nucleare si dovrà porre il problema delle materie prime. Quanto sta accadendo in Niger, uno dei maggiori produttori di uranio, e in generale nei Paesi africani che, nel volgere di pochi anni, sono passati sotto l'influenza cinese o, peggio, russa ci deve ammonire circa il rischio da dipendenza da potenze globali in ordine all'approvvigionamento delle materie prime. La rivoluzione energetica deve passare quindi anche da un nuovo e più attento presidio geopolitico delle catene di approvvigionamento. Di questo si dovranno certamente far carico negli anni a venire il vice *premier* e ministro degli esteri Tajani e il ministro della difesa Crosetto, ma certamente siamo in buone mani.

Ministro, i recenti fatti di Palermo e Caivano hanno accresciuto l'attenzione sul problema, già noto, dell'esposizione dei minori a contenuti pornografici e violenti mediante soprattutto i collegamenti in Rete. Con l'inizio della pandemia si è assistito all'adozione di strumenti normativi a livello internazionale e sovranazionale dedicati ai diritti delle persone di minore età nell'ambiente digitale, volti a prevenire e contrastare l'abuso e lo sfruttamento sessuale *online* di minori, incluse la pornografia minorile e la pedopornografia. La novità più rilevante in questo ambito è la proposta di regolamento della Commissione europea dell'11 maggio 2022, che prevede tra l'altro la creazione di un centro europeo per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento e dell'abuso sessuale dei minori, che muove da analoghe esperienze canadesi e australiane. Il futuro regolamento, se approvato, sostituirà il regolamento UE del 14 luglio 2021, n. 1232, il cosiddetto regolamento *chat control*. La questione relativa all'accesso, da parte di minorenni, a materiale pornografico è menzionato nel commento generale n. 25 sui diritti dei minorenni in relazione all'ambiente digitale, adottato nel 2021 dal Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che incoraggia gli Stati a proteggere i minorenni da contenuti dannosi e inattendibili, e garantire che le imprese e altri fornitori di contenuti digitali sviluppino

Da tempo sono disponibili sul mercato strumenti fruibili in grado di monitorare ed eventualmente regolare la navigazione in Rete dei minori, il principale dei quali è il cosiddetto *parental control*, la cui diffusione è però limitata. Recentemente è stato adottato il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, che include la sicurezza dei minori in ambito digitale, volta a diffondere l'uso del *parental control* con relative campagne informative. vorrei quindi chiederle di sapere quali siano le iniziative del Dipartimento per le politiche della famiglia in relazione all'alfabetizzazione digitale e mediatica, a tutela dei minori e alle campagne informative di cui l'articolo 14 del decreto-legge del 15 settembre 2023, n. 123, fa parte. PRESIDENTE.

Signor Presidente, ringrazio gli interroganti per aver posto questo quesito, che purtroppo è molto attuale. L'esposizione dei minori a contenuti pornografici e violenti è considerata sempre più, anche a livello internazionale, un problema di salute pubblica, in quanto può compromettere il loro sviluppo psicofisico e il loro benessere, considerando, fra l'altro, che l'età media di accesso ai siti con questi contenuti è sempre più precoce ed arriva ormai a sei o sette È un tema che abbiamo affrontato fin dall'inizio dell'attività di Governo, in realtà senza aspettare di essere sollecitati dai drammatici casi di cronaca cui abbiamo assistito. Infatti, nella scorsa legge di bilancio abbiamo stanziato tre milioni di euro per il biennio 2023/2025 per la promozione di progetti educativi di alfabetizzazione mediatica e digitale a tutela dei minori. A giugno sono stati poi definiti i criteri e le modalità di attuazione di questa iniziativa. Dopo però gli avvenimenti di Palermo e Caivano, il Governo ha stabilito di incrementare le tutele con ulteriori misure. Uno dei mezzi principali per impedire che la fruizione della rete da parte dei minori sia incontrollata è appunto il cosiddetto *parental control*. Si tratta di strumenti come applicazioni, *software* e soluzioni di rete che possono escludere l'accesso a siti ritenuti non adeguati dai genitori, regolare anche i tempi di accesso alla rete e comunque monitorare la navigazione del minore. Sono soluzioni tecnologiche già disponibili da tempo e anche molto efficaci, in particolare per evitare che i più piccoli possano incappare casualmente in contenuti inadeguati e, e, in genere, per educare da subito a un uso consapevole di Internet. I genitori possono avvalersene adattandole all'età e alla maturità dei propri figli: non una censura, quindi, ma uno strumento educativo in mano alle famiglie, che però è stato fin qui molto poco utilizzato, come giustamente sottolineato dai senatori interroganti. Nel cosiddetto decreto Caivano abbiamo quindi previsto che, entro un anno, i produttori assicurino, all'atto dell'immissione sul mercato dei dispositivi di comunicazione elettronica, che i sistemi operativi installati

produttori dovranno obbligatoriamente inserire nelle confezioni di vendita di ogni dispositivo elettronico. Avvalendoci anche delle competenze dell'Agcom, elaboreremo poi linee guida specifiche sull'uso del *parental control*, rivolte ai genitori e agli educatori in generale, ma anche agli stessi minori, che pure saranno disponibili sul nostro sito istituzionale. È necessario però che anche sul territorio vi siano presidi cui le famiglie possano facilmente rivolgersi per informazioni, consulenze e servizi di alfabetizzazione digitale. Sempre con il decreto citato, abbiamo affidato questo compito ai centri per la famiglia già esistenti e finanziati tramite il fondo per le politiche per la famiglia, ai quali, per la prima volta, viene attribuito un compito specifico per legge. Anche questa, io ritengo sia un'innovazione positiva.

e ha sottolineato l'impegno del Governo su un tema che ci affligge tutti: genitori, nonni e figli. Questo infatti è un tema che comunque, ad oggi, è diventato di primaria importanza. Conosciamo l'impegno economico, che lei prima ha raccontato con i numeri, e sappiamo anche dell'impegno fattivo sul territorio, quindi ci sentiamo soddisfatti della sua risposta, di cui la ringrazio.